e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale

nella seduta pomeridiana del 9 luglio si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo. Prima di passare all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati, avverto che gli ordini del giorno presentati, avverto che gli ordini del giorno G102 e G103 saranno esaminati prima della votazione dell'articolo 2.

l'ordine del giorno G100 fa riferimento ad una modificazione apportata dalla Commissione.

vuole escludere qualsiasi tipo di interferenza del Comitato parlamentare, il parere è favorevole, ove si addivenga ad una riformulazione che prenda atto delle affermazioni del ministro Quagliariello, impegnando quindi il Governo a far concludere l'attività della Commissione prima dell'avvio dell'esame dei disegni di legge.

del giorno G106 prevede che «la riforma costituzionale sia in primo luogo finalizzata ad un ridimensionamento dei costi della politica». Il parere è favorevole se si accetta la seguente riformulazione: «la riforma costituzionale sia finalizzata anche ad un ridimensionamento dei costi della politica». Sull'ordine del giorno G109, come i colleghi sanno, è nel frattempo intervenuto il disegno di legge del Governo.

all'ordine del giorno G110, sarebbe forse meglio parlare di una «razionalizzazione delle competenze tra i diversi livelli di governo». G111 il parere è favorevole se il testo si ferma alla parola «Regioni».

Senatore Calderoli, dicevo di mettere un punto dopo la parola «Regioni». Siccome stiamo parlando di Statuti speciali, è assolutamente ovvio che stiamo parlando di Regioni autonome, quindi va benissimo anche la riformulazione del Governo, non ho alcuna difficoltà. Mi pareva che la formulazione fosse assolutamente ridondante visto che il riferimento agli Statuti speciali già definisce l'ambito

prima dell'avvio evitando qualsiasi tipo di interferenza che possa limitare l'autonomia del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato approva.**

in quanto siamo preoccupati di questo procedere in deroga e per urgenza e siamo preoccupati di essere così soli ad essere preoccupati. E siamo preoccupati di sentire da Enrico Letta il 5 giugno 2013 dire: «Ciò che stiamo facendo è dovuto ad uno stato di eccezione». Stato di eccezione o stato di necessità? Bisogna stare attenti alle parole e ai *lapsus* eventuali. Quale stato di eccezione voleva indicare il *Premier*? Cos'è lo stato di eccezione? Lo Stato di eccezione, signori, è uno dei concetti chiave dell'ontologia politica di Carl Schmitt, contrapposto allo Stato di diritto, in quanto si configura, appunto, come una situazione in cui il diritto è sospeso, i tre poteri fondamentali unificati. Non voglio forzare il ragionamento ricordando chi e quando utilizzò lo stato di eccezione come soggetto politico che pretende per sé il controllo totale in ogni ambito della società: lungi da me. Ma signori, bisogna stare attenti alle parole, soprattutto in questi anni difficili di continuo e sistematico attacco alla centralità del Parlamento, di attacchi alla magistratura, di procedure d'urgenza, di riforme costituzionali. Sono orgogliosa, signori, di essere dalla parte di chi in queste Aule porta indefessamente il diritto di esistenza, di resistenza dei cittadini che sono fuori, spesso senza parola.

presentato all'articolo 1 seguono tutti quanti un criterio che noi abbiamo varie volte illustrato, e tra l'altro posto nella discussione generale, in tutti gli interventi che sono stati fatti da parte del mio Gruppo.

non pensiamo assolutamente che tra l'altro anche modifiche che evidentemente questo Comitato che la maggioranza ambisce a fare per ciò che attiene alle forme di elezione del Presidente della repubblica, debbano di per sé portare ad un certo tipo di sistema elettorale.

provare anche a recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini, le istituzioni e

Invito tutti quanti a riflettere: avete il coraggio, visto anche quello che è accaduto ieri, di far rischiare al Paese di tornare alle elezioni ancora con il "Porcellum"?

È una delle questioni che purtroppo, ahimè, come un po' tutti i nostri emendamenti nell'ambito del lavoro della Commissione affari costituzionali, non sono state

del criterio di proporzionalità all'interno del Comitato, che, a nostro avviso, non è rispettato. Questo è un altro *vulnus*, noi avevamo chiesto che fosse garantita la rappresentanza di tutti i Gruppi presenti sia alla Camera che al Senato, sempre con l'argomento che il Senato ancora non l'abbiamo abolito

preciso, e che abbiamo sottoposto costantemente all'attenzione della Commissione riguarda questa ossessione del cronoprogramma,

l'1.109. Noi non riteniamo - è una delle questioni che abbiamo sempre posto con una certa evidenza - di dover scandire in modo così preciso

state accolte e neanche lontanamente considerate, pongo nuovamente all'attenzione dell'Aula tale questione, che è certamente delicata, ma è certamente degna

con l'emendamento 1.150, sin dalla sua presentazione in Commissione, intendevo fornire un elemento di completezza al Comitato ed ai suoi componenti e quindi una volontà di partecipare. Consapevole della criticità che tale modifica comporta e soprattutto alla luce delle sollecitazioni che mi sono state poste, ho però ritenuto di doverlo ritirare anche per evitare una sua inutile bocciatura.

il mio vuole essere un gesto di responsabilità, ma nello stesso tempo di sana provocazione, anche per far capire che noi eletti all'estero ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo quando si tratta di avviare procedimenti legislativi delicati e complessi, partecipando attivamente all'urgente ed improrogabile stagione di riforme di cui il nostro Paese ha bisogno. Infatti, oltre alla presenza, garantita dalla norma, di un componente del Gruppo e di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche che ritengo assolutamente condivisibile e doveroso - sarebbe stato il caso di garantire la presenza di un parlamentare eletto nella circoscrizione Estero, al fine di consentire un opportuno equilibrio di rappresentanze all'interno del Comitato, la cui straordinarietà di responsabilità costituzionale, in un momento delicato sotto il profilo sociale e politico, non potevano esimere dal coinvolgere una platea parlamentare e dunque elettorale complessa e distinta. La sua specificità non soltanto è legittimata da dinamiche elettorali distinte rispetto a quelle vigenti sul territorio nazionale, ma soprattutto dalla sussistenza di specifiche tematiche e progettualità affrontate dal Comitato, anche perché queste richiederanno approfondimenti che potranno essere avviati soltanto con un parlamentare eletto nella circoscrizione Estero. Pertanto, con questo mio gesto di buonsenso e di responsabilità ritengo opportuno rivolgere all'Assemblea del Senato ed ai Gruppi parlamentari che saranno chiamati a delineare la composizione del Comitato un invito a garantire la presenza di un rappresentante della circoscrizione Estero, proprio per assicurare la dovuta legittimità alla composizione del Comitato *in fieri*. Sarà mia cura, dunque, ritirare l'emendamento 1.150 (così come 2) in ragione dell'opportunità politica correlata allo stesso e provvederò a trasformarlo, signor Ministro, in un ordine del giorno che raccolga comunque lo spirito delle proposte emendative originarie. Non abbiamo condizionamenti da porre né pressioni; il nostro vuole essere un invito al buonsenso.

tende a riportare a 40 il numero dei membri del Comitato, aumentati a 42 con l'emendamento approvato dalla 1a Commissione che ha indicato i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali come membri di diritto.

Presidente, proprio per rispondere alle osservazioni che anche da ultimo sono venute dai colleghi intervenuti nell'illustrazione degli emendamenti,

Voglio ricordare ancora che abbiamo teso ad integrare il testo prevedendo la presenza dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari in sede di programmazione dei lavori, coerentemente a quanto previsto dai Regolamenti del Senato e della Camera

al fine di evitare problemi di ordine interpretativo, stante l'accezione che potrebbe sottendere impropriamente il riferirsi a una consistenza numerica complessiva dei Gruppi di Camera e Senato.

Immaginiamo che possano partecipare a tale consultazione, che prevediamo davvero ampia, i cittadini maggiori di sedici anni, anche nella considerazione che saranno quelli che per più tempo potrebbero vedere gli effetti di tali modifiche costituzionali.

finché i cittadini non abbiano avuto modo di esprimersi su di esso, in modo tale da aver compiutamente idea di quale sia il ricevimento il ricevimento degli eventuali interventi sulla Costituzione in quell'ambito. Riteniamo, infatti, che i precedenti tentativi di riforma della nostra Costituzione non abbiano avuto esito felice in tantissimi casi appunto per la distanza tra il corpo elettorale, ossia i cittadini,

mantiene la riduzione da quattro a due dei Segretari. Esso inoltre interviene poi su un aspetto che riteniamo molto importante: il criterio di elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza qualora, a seguito delle votazioni si raggiungano situazioni in cui i due candidati ottengano lo stesso numero di voti. Ebbene, in questo caso l'emendamento sostituisce il criterio dell'anzianità con quello della giovinezza.

In caso di assenza dalle sedute del Comitato ai componenti sarà ritenuto un trentesimo della componente variabile della diaria per ogni giornata». È un emendamento che definisco del buonsenso e della normalità: infatti che, se si è assenti, venga trattenuta parte della diaria. In luogo di un'impropria disciplina incidente sul numero legale delle Assemblee, con l'emendamento si intende applicare al Comitato il regime delle trattenute per i senatori assenti dalle Commissioni permanenti previsto con delibera del Consiglio di Presidenza del Senato del 14 dicembre 2011.

di sostituire, anche temporaneamente, un membro del Comitato impossibilitato a partecipare ai lavori o ad una seduta. Il divieto incide sui Gruppi minori e di opposizione e, se ha un senso nelle Commissioni di inchiesta, che svolgono un ruolo simile a quello di un collegio giudicante, non ha invece alcuna ragione d'essere in una Commissione referente.

che l'emendamento intende sopprimere, riguarda la valenza e il rapporto tra le fonti dell'ordinamento. In particolare, la disciplina che regola il numero legale nelle Assemblee di Camera e Senato è sancita dai rispettivi Regolamenti parlamentari,

ancorché adottata con legge costituzionale. Peraltro, pur private di molte competenze, le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato continueranno ad operare e non sarà quindi agevole seguirne i lavori

l'equivoco o l'ambiguità cui alludeva la collega De Petris francamente è da escludere totalmente: si parla esclusivamente delle leggi elettorali conseguenti alle eventuali riforme costituzionali

all'emendamento 1.103, la senatrice De Petris ha posto la questione della composizione proporzionale e della presenza di tutte le rappresentanze parlamentari. che il criterio misto, adottato nel disegno di legge, incide esattamente su una questione molto seria ai fini della definizione della proporzionalità. riferisco al fatto che, trattandosi di comitato paritetico, comprendente rappresentanti dell'una e dell'altra Camera, qualora avessimo adottato, o adottassimo, esclusivamente un criterio proporzionale,

essendo stato applicato il premio di maggioranza nella definizione dei risultati elettorali, è chiaro che ci troviamo in una condizione nella quale il Comitato non rappresenterebbe

disegno di legge assicura in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo, con ciò riferendosi a ciascun Gruppo presente alla Camera e/o al Senato. Tutti sappiamo che ci sono Gruppi costituiti presso una Camera, che non sono costituiti presso l'altro ramo del Parlamento. L'emendamento della senatrice De Petris, che vorrebbe la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo presente sia alla Camera che al Senato, potrebbe essere interpretato nel senso che verranno rappresentati esclusivamente quei Gruppi che abbiano rappresentanza sia alla Camera che al Senato. Ritengo, quindi, che la formulazione scelta dalla Commissione sia più rispettosa degli stessi principi di cui la senatrice De Petris

che il numero dei Segretari è già stato ridotto a due, proprio in accoglimento di una richiesta del Movimento 5 Stelle, e che il criterio del più giovane di età è un criterio che non rintracciamo mai nei Regolamenti parlamentari. Capisco il punto di principio, ma penso anche che sarebbe estremamente penalizzante per i senatori poiché l'età anagrafica

1.111, per le ragioni che dicevo prima circa la presenza di tutti i Gruppi alle sedute di programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza. Il parere

che così riscriverebbe il dispositivo: «si impegna a prevedere che i criteri applicativi, di cui al primo periodo, comma secondo, dell'articolo 1 siano definiti al fine di garantire la più ampia rappresentanza dei Gruppi parlamentari».

l'emendamento 1.101 in particolare andrebbe ad affrontare la questione legata ad eventuali voti di maggioranza all'interno del Comitato. Ricordiamo che i due Presidenti che si aggiungono ai quaranta membri fanno parte della maggioranza. Quindi, invito tutti a tenere in considerazione questo aspetto.

si fa un riferimento al Governo. A me sembra inverosimile che si faccia riferimento a un qualunque tipo di ruolo del Governo quando si dovranno nominare i membri del Comitato mettendoci all'interno un eletto all'estero. Francamente non riesco a capire cosa c'entri il Governo.

che chiede al Governo una interlocuzione, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, a me pare che la risposta del Governo non avrebbe potuto essere differente. È evidente che quei limiti

Signor Presidente, a questo punto, visto che ho avuto l'opportunità di leggere l'ordine del giorno G1.150, vorrei leggerlo anche all'Assemblea. Il dispositivo recita: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità,

Presidente, però mi preoccupa il passaggio successivo, là dove recita: «eventualmente attraverso il coinvolgimento del Comitato per le questioni degli italiani nel mondo istituito presso il Senato della Repubblica, segnatamente per quanto riguarda il procedimento legislativo relativo alla riforma della legge elettorale».

in quanto è una novità il trattamento speciale riservato agli eletti all'estero, mentre è ben diverso, come nella precedente formulazione dell'emendamento, farlo seguire alla tutela delle minoranze linguistiche, che

tutti i Gruppi presenti in entrambe le Camere - discussione che abbiamo fatto fino a due minuti fa - e garantire la rappresentanza degli eletti all'estero, che comunque in questo Parlamento siedono, essendo iscritti ai Gruppi

mi sono preoccupato nell'ascoltare il presidente Calderoli, perché ne conosco la raffinata arguzia e l'intelligenza politica e ho visto il testo dell'ordine del giorno Francamente, nessuno espropria nessun altro: semplicemente i colleghi eletti all'estero - perché questa è la realtà - si sono preoccupati di essere coinvolti nell'elaborazione di un'eventuale disciplina nuova che riguarderà anche loro come eletti all'estero. La preoccupazione è condivisibile: se fossi un eletto all'estero avrei esattamente la stessa preoccupazione.

del giorno G1.150. Se poi vogliamo riformularlo, possiamo farlo, ma lo spirito è questo. Peraltro, ciascuno di noi, anche nel valutare la possibilità di una revisione della normativa attuale degli eletti all'estero, ha tutto l'interesse a non dare un cattivo segnale agli italiani residenti all'estero. Non è che abbiamo scherzato: prima li abbiamo associati al processo legislativo facendoli eleggere all'estero, oggi non li vogliamo neanche associare nella discussione su un'eventuale modifica di questa disciplina. Ritengo quindi che l'ordine del giorno

parte del Comitato tutti i Gruppi: tutti i Gruppi, lo dice il testo e non un'interpretazione libera. Mi pare che lo spirito autentico fosse quello di dire poiché il Governo presenterà disegni di legge in materia di revisione costituzionale e, tra questi disegni di legge, potrebbe anche accadere che ci fosse, qualora approvata, una legge elettorale ad essi conseguente, i senatori e i deputati eletti all'estero chiedono un confronto con il Governo. L'elemento di ambiguità è dato dalle parole «un confronto attivo e costante del Comitato *in* *fieri*»: il Comitato è parlamentare e avrà cura di mantenere il contatto con i colleghi eletti all'estero. Questo impegno è rivolto al Governo e, quindi, nella fase non parlamentare, ma, come diceva il ministro Quagliariello,

quale la stessa ha paventato un rischio di discriminazione dell'Assemblea del Senato per la questione dell'età anagrafica rispetto ai colleghi della Camera, vorrei sommessamente farle notare che tale rischio non sussiste, in quanto lo stesso emendamento prevede che la composizione dell'Ufficio di Presidenza sia ugualmente distribuita

Mi sembra un modo sano e valido per legare il lavoro fatto all'interno delle istituzioni a quello che avviene nel mondo normale: se non vai a lavorare, non vieni retribuito per quella giornata di lavoro. invito, in maniera serena e costruttiva, a rivedere se possibile il parere, invitando ad un accoglimento di questo emendamento. Ne

e. Se così dovesse essere, procediamo al ritiro della tessera. C'è un eccesso di luminosità sospetto in quella zona.

ringrazio, signor Presidente.

l'Assemblea costituente nacque il 25 giugno 1946 e terminò il 31 gennaio 1948 e fu composta da

Ci preoccupa anche perché - come noto - esprimiamo un dissenso molto forte e netto rispetto all'ipotesi di quello che secondo noi è un vero e proprio stravolgimento dello spirito della Carta costituzionale. Noi difendiamo fortemente la Repubblica parlamentare e siamo radicalmente contrari a qualunque forma di presidenzialismo e anche di semipresidenzialismo.

proprio nei giorni successivi all'elezione del presidente Napolitano. Vi chiederete cosa c'entra tutto questo, ma in realtà c'entra moltissimo. Infatti, l'attuale Presidente del Consiglio, l'onorevole Letta,

(chiedo alla presidente Finocchiaro di ascoltare e, magari, di interloquire su questo punto, perché il suo parere mi interessa sempre): viviamo in una fase in cui da parte dell'opinione pubblica generale della popolazione di questo Paese, anche alla luce della crisi della politica, arriva una fortissima richiesta di partecipazione. Si è parlato moltissimo di democrazia partecipativa, partecipativa, della necessità di introdurre nella Costituzione strumenti di rafforzamento degli istituti della democrazia diretta

- molto differentemente da quanto accade in altre democrazie del mondo dove esistono sistemi presidenziali e semipresidenziali, ma esistono anche i contrappesi

i meccanismi istituzionali per temperare il potere politico dell'eventuale uomo solo al comando, ci si chiede: è compatibile l'uomo solo al comando con l'idea di allargamento della base della democrazia partecipativa e con la richiesta forte che viene da ampi settori della popolazione italiana che chiede maggiore coinvolgimento e maggiore possibilità di incidere sui processi reali?

della nostra Costituzione e della nostra Repubblica trasformando la Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale, la componente SEL del Gruppo Misto (ma io penso insieme a noi anche diversi milioni di italiani) difenderà in tutti i modi la democrazia parlamentare tentando di impedire questa deriva. *(Applausi

la ricostruzione di un forte rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, l'efficienza del sistema democratico senza manomettere l'impianto

in esame mira a stabilire che ulteriori disposizioni riguardanti il Comitato debbano essere esclusivamente di natura organizzativa.

perché il tutto sia il più possibile trasparente, sempre, e chiaro. Chiederemo anche (quindi ribadiamo questa nostra volontà) che il voto sia sempre nominale, che sia sempre possibile risalire - e un sistema elettronico è l'unico che lo consente - a «chi ha votato cosa», crediamo sia fondamentale che i cittadini sappiano «chi ha votato cosa», sì, no o astenuto, per ogni singolo emendamento, sia in Commissione, sia in Aula.

materia elettorale, dato proprio il dibattito in atto da tempo tra tutte le forze politiche e le esperienze delle ultime competizioni elettorali, che hanno mostrato una crescente disaffezione

il rispetto del principio di rappresentatività democratica, in modo che agli elettori sia garantita la possibilità di scelta degli eletti, e la garanzia delle imprescindibili esigenze di governabilità. Pertanto, auspico che l'intera Assemblea e tutte le forze politiche, che a parole si dicono favorevoli al

oltre che incrementare il fondamentale principio della pubblicità dei lavori in seno al Comitato attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito Internet del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali a disposizione del pubblico e della stampa. Tale proposta modificativa segue il solco della Costituzione (articolo 64), da cui è sotteso che un sistema di democrazia parlamentare veda l'azione pubblica come regola e il segreto, invece, come anche perché il procedimento decisionale muta significativamente in una sede pubblica o segreta. Signor Presidente, gli italiani con questo disegno di legge al tentativo di esternalizzare ad un'emanazione governativa la formulazione di un indirizzo che non dovrebbe vedere invece estraneo, o relegato in posizione subalterna, il Parlamento. Non si può dunque pensare che il cosiddetto Comitato che questi indirizzi dovrebbe poi ponderare e sviluppare sia dispensato dal dovere di trasparenza sul proprio operato, sottraendo al popolo la piena formazione del giudizio non solo sulle soluzioni che lor signori vorranno calarci, ma anche sulla natura e sulla qualità del dibattito. caso infatti - badate bene - sarebbe ancor più difficile smentire il dubbio che tali soluzioni siano predeterminate: solo formalmente sviluppate nella sede dichiarata e stabilite invece altrove, e per una incombente committenza.

questo è un articolo molto importante, perché riguarda la modalità dei lavori delle Assemblee,

E qui arrivo al punto per noi dirimente e più delicato, che riguarda il diritto dei parlamentari, di ogni singolo deputato e senatore.

la centralità del Parlamento è fondamentale, e quindi non può esservi equiparazione. Proprio perché vi dovrebbe essere

della presentazione di emendamenti da parte, ad esempio, dei relatori, ogni singolo senatore può presentare subemendamenti, con l'attuale articolo 3 ciò sarà impedito, perché sarà concesso subemendare solo ed unicamente ad un Presidente di Gruppo,

L'emendamento, in subordine al precedente, prevede il sottocomitato, ma non la procedura emendativa straordinaria. Al comma 3 si prevede l'applicazione senza varianti dei Regolamenti di Camera e Senato e s'inserisce nel sottocomitato il relatore di minoranza.

astrattamente all'inizio dell'esame: una forzatura inopportuna in materia delicata come quella costituzionale.

del dibattito politico e del rischio concreto che le contraddizioni aperte oggi rispetto al Governo delle larghe intese possano far tornare il Paese al voto in tempi più rapidi di quelli previsti. Noi pensiamo che occorra costruire un meccanismo che consenta al Paese di avere una clausola di salvaguardia: se si dovesse tornare al voto non si può più farlo con la legge "porcellum". quindi che sia un errore questa equiparazione della legge elettorale alla forma di Governo e alla riforma costituzionale. Peraltro, non ci convince per niente nemmeno la tesi secondo la quale ad ogni forma di Governo corrisponde necessariamente una legge elettorale,

esplicito: il Comitato tratterà soltanto i progetti di legge ordinaria di riforma di sistemi elettorali che siano conseguenti e coerenti (su questo c'è stata una discussione) con il progetto di riforma. Per quanto riguarda i progetti di legge elettorale dove questa correlazione non c'è, oggi, domani, la funzione referente rimane alla Commissione affari costituzionali. Noi possiamo (e, dal nostro punto di vista, è auspicabile che lo si faccia rapidamente) trattare subito, nelle more della revisione costituzionale, la possibilità di modificare la legge elettorale vigente per le Camere in maniera transitoria: subito. Il progetto in corso non mette in discussione questa possibilità. Quindi ci sono due strade: una, che è affidata al Comitato, è quella di disciplinare anche la legge elettorale conformemente, coerentemente e conseguentemente al progetto di riforma; ma non c'è dubbio che oggi e domani il Parlamento, la Commissione affari costituzionali possano transitoriamente mettere mano alla legge elettorale, come noi auspichiamo.

prendo la parola anche se non ce ne sarebbe bisogno, perché la situazione è chiarissima, soprattutto dopo l'emendamento della relatrice

della modifica della legge elettorale a prescindere dal Comitato e da quello di cui stiamo discutendo oggi. Ci sembra quindi eccessivo che si ritorni su argomenti che sono e ribadisco il concetto (perché chi ci ascolta potrebbe fraintendere) che il Gruppo che io rappresento in questo momento è assolutamente favorevole alla trattazione di questo argomento in Commissione ed in Aula e lavorerà in tal senso,

che «La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento,

Come ricordato dalla senatrice Nugnes, noi siamo preoccupati per questo modo di procedere sempre in deroga e per urgenza e siamo ancora più preoccupati di essere i soli ad essere preoccupati

riducendo la sperequazione rispetto alla tempistica concessa al Governo. L'emendamento 3.20 parifica i parlamentari ed il Governo nei termini emendativi, non essendoci ragione alcuna per attribuire vantaggi all'Esecutivo. 3.21 integra il testo con criteri di emendabilità già stabiliti dal Regolamento.

da parte del Partito Democratico, perché si cominci immediatamente, in sede di 1ª Commissione, a discutere i disegni di legge tendenti ad abrogare il «porcellum». La questione che abbiamo posto è che l'aver inserito e l'aver voluto insistere nell'inserire la materia elettorale conseguente alle modifiche all'interno del lavoro del del Comitato è in qualche modo, a nostro avviso, onestamente non spiegabile attraverso il fatto che poi debba essere messo tutto quanto a regime. Vi farò omaggio

il doppio turno alla francese ‑ comporterà immediatamente l'adozione del doppio turno alla francese (e potrei fare anche altri esempi): non è esattamente così.

Il caso si può porre ad esempio nel momento dell'eliminazione del Senato, che è uno degli obiettivi; ma lì l'adeguamento sarebbe anche abbastanza semplice.

irragionevole a nostro avviso, data la delicatezza della materia e la presenza di un termine finale di deliberazione, con un meccanismo meno penalizzante per i singoli parlamentari, in modo da tutelare anche quelli dissenzienti dai Gruppi,

ho votato la parte in cui correttamente si recupera la possibilità di partecipazione al processo costituente consentendo

tutto il processo costruito (che già rappresenta una deroga all'attuale sistema di revisione costituzionale) senza possibilità di partecipazione effettiva.

ringrazio il senatore Caliendo per l'intervento testé svolto. Magari avrebbe fatto meglio ad appoggiare nelle passate votazioni qualche nostro emendamento che andava esattamente in questa direzione; comunque, meglio tardi che mai. Dunque, condivido il suo intervento e i rilievi che egli ha formulato, perché attengono esattamente a un tema sul quale stiamo battendo da moltissimi giorni, cioè la centralità del Parlamento la possibilità per tutti i parlamentari, per le opposizioni, per quelli che sono in dissenso dai Gruppi e per ciascuno di noi, di fornire il proprio contributo a tale processo.

ho sentito in Aula uno splendido intervento che all'epoca condivisi molto sul tema del mandato imperativo e, in realtà, ha molto a che fare questo tema con il mandato imperativo.

che quell'articolo della Costituzione non esista

Vorrei ricordare al senatore Caliendo che, mentre che quello che dice è assolutamente vero per la Commissione dei 75 (quindi il corrispondente all'attuale Comitato), non credo sia vero, invece, circa il regime di emendabilità del testo elaborato dalla Commissione dei 75 da parte dell'Aula. Vorrei anche ricordare che ci troviamo in un sistema nel quale, sia pure con una limitazione che riguarda i subemendamenti agli emendamenti del Comitato e del Governo (limitazione che poi dà la possibilità di presentare subemendamenti ai Presidenti di Gruppo, a dieci senatori o a venti deputati mantenendo un'ordinarietà nella possibilità di presentare subemendamenti), la storia dei Regolamenti di Camera e Senato

attraverso le forme proprie, la possibilità di intervenire sul testo evitando, dall'altra parte, che attraverso queste modalità si mettano in opera meccanismi ostruzionistici che impediscano il fisiologico fisiologico svolgersi del rapporto tra maggioranze (non maggioranza di Governo) e opposizioni all'interno delle Aule parlamentari. Questo è il criterio al quale ci siamo attenuti. Voglio ricordare a tutti i colleghi che non è affatto vero che ciascun componente dell'Assemblea non ha la possibilità di presentare emendamenti. È assolutamente chiaro, infatti, che fino a cinque giorni prima i componenti dell'Assemblea possono ripresentare emendamenti respinti dal Comitato o presentare emendamenti al testo del Comitato, ovviamente in diretta correlazione con le parti della Costituzione modificate. A questo aggiungo che c'è un'ulteriore tema sul quale il Comitato si è soffermato (perdonatemi se vi trattengo sulla questione, ma è molto seria) ed è il fatto che da una parte, ovviamente, ci deve essere la facoltà-potere di presentare emendamenti, ma dall'altra parte trovo che bisogna tutelare allo stesso modo il diritto di ciascuno dei componenti dell'Aula di conoscere, studiare e poter compiutamente apprezzare il contenuto di ciascun emendamento. una scansione temporale che consenta in ogni momento la presentazione di emendamenti ma non dia all'Aula e a ciascun componente la possibilità di riflettere sul contenuto e sulle conseguenze di ciascun emendamento

che possono essere contestate. Voglio, però, rassicurare i colleghi che avvertendo la forza dei loro suggerimenti e il contemperamento con le esigenze di cui abbiamo parlato questo è stato condiviso dalla maggioranza della Commissione come l'assetto più equilibrato. all'emendabilità dei testi esistono coerentemente e sono previste dai Regolamenti di Camera e Senato per particolari materie. materie. Inoltre, quando si è andati - per esempio - con la Commissione bicamerale D'Alema a definire l'ambito delle possibilità, l'emendabilità del testo in Aula

anche per la presentazione dei subemendamenti. Noi riteniamo che alla stregua di questa prescrizione i Gruppi di minoranza non siano sufficientemente tutelati. Ora, facendo seguito a svariati appelli del Capo dello Stato, dei quali i colleghi conoscono sicuramente il contenuto, nei quali è stato espresso l'auspicio che le riforme siano per la maggior parte condivise da tutte le Assemblee,

non so se sarà efficace. A maggior ragione, proprio perché vi è stata questa forte equiparazione, incongrua,

Non vi sono giustificazioni legate alla procedura, ché anzi la procedura di revisione costituzionale ci dovrebbe imporre di riconoscere a tutti

vi siete fatti tutti una vaccinazione di garanzia, che vi assicura di trovare sempre le soluzioni più adeguate e che non intervengano

Se queste sono le premesse, credo - anzi, sono convinto - che tutto il lavoro che verrà fatto in questo Comitato sarà quello che vorranno fare i due partiti che sostengono la maggioranza di Governo. Quindi mi ricollego a quanto è stato detto da altri colleghi: non vedo la volontà di avere una maggioranza che deve essere la più ampia possibile proprio quando andiamo a toccare la nostra Costituzione. Come tanti emendamenti di buonsenso, anche il 3.30 è semplicissimo. Esso prevede, al fine di favorire la subemendabilità nei brevi termini concessi, la redazione di una relazione illustrativa degli emendamenti del Governo, tenuto anche conto del fatto che esso non deve rispettare termini di deposito altrettanto stringenti quanto quelli previsti per i parlamentari di maggioranza e di opposizione.

altri emendamenti che tentano di espungere dal testo gli elementi assolutamente incongrui.

che nel dibattito che si è svolto prima dell'approvazione delle mozioni, in quest'Aula come nell'Aula della Camera la mia parte politica disse in modo molto esplicito che speravamo - lei, Ministro, lo sa bene

quello che non ci saremmo augurati, cioè che invece il processo di riforme costituzionali era solo e unicamente un affare della maggioranza.

4. L'emendamento comporterebbe l'eliminazione della tempistica speciale per i lavori del Comitato e conseguentemente l'applicazione della procedura regolamentare ordinaria. Per meglio farvi comprendere l'importanza di questo emendamento, vorrei ricordare un appello di un nostro Padre costituente: un appello accorato di Piero Calamandrei nel discorso ai giovani tenuto alla Società umanitaria nel gennaio del 1955. Ve lo voglio ricordare, anche se siete un po' distratti: si parla di Costituzione qui, non stiamo parlando di argomenti molto leggeri! M5S)*. Piero Calamandrei, nel 1955, ci mandava un accorato appello e diceva ai giovani dell'epoca: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione». Ora, mentre uno dei nostri grandi Padri costituenti ci ha lasciato questo meraviglioso invito a una sommessa meditazione sulla nostra Carta costituzionale, qui cerchiamo di imporre una tempistica speciale, accelerata, svilente. La soppressione dell'articolo 4 è necessaria per evitare il solito malcostume di mescolare le carte e creare confusione. I Padri costituenti hanno impiegato molto tempo per concepire la nostra Carta costituzionale e hanno anche stabilito una tempistica per la sua modifica, mentre qui vogliamo stabilire tempistiche veramente ridicole, tempistiche che non consentono la dovuta trasparenza e anzi alimentano una fretta che porterebbe ad atti potenzialmente zoppi e inefficienti. Non si parla qui di una singola modifica, facciamo attenzione, ma di infiniti disegni di legge. Troviamo quindi svilente asservire la nostra meravigliosa Carta costituzionale a tempi che non sono quelli del popolo. Il popolo non chiede di avere fretta nel cambiare la Costituzione, chiede con urgenza di occuparsi della sua disperata condizione di vita. *(Vivi

raccontano di una volontà difficilmente perseguibile in ragione delle condizioni politiche di questa anomala maggioranza, con l'idea di colpire, attraverso una costruzione organica degli interventi sulla Parte II della Costituzione, tutte le leggi costituzionali che quei contenuti richiamano, ad iniziare dagli Statuti speciali delle Regioni. Mi riferisco in modo particolare a quelli della Sicilia e della Sardegna che nascono con leggi costituzionali, al momento più direttamente connesse alla fase costituente. Nell'idea, esplicitata nel contenuto di questo provvedimento, di connettere direttamente la trasformazione della nostra Costituzione, soprattutto per quanto attiene alla parte relativa alla forma di Governo, con l'individuazione di coerenti progetti di legge, vediamo una volontà autoritaria e accentratrice rigettata dalla Parte I della Costituzione, la parte intoccabile, ma è soprattutto rigettata dalla parte che contiene i principi fondamentali.

riteniamo che l'emendamento in votazione ponga una questione ineludibile e che probabilmente sia stata una svista non aver inserito un inciso che specificasse il fatto che i lavori del Comitato sono pubblici. Se ci pensiamo, ancora oggi possiamo comprendere con maggiore nettezza alcuni passaggi della nostra Costituzione perché possiamo rileggere i resoconti e i verbali della Costituente. Certamente, all'epoca non esisteva la possibilità di rendere pubblici tali lavori, a meno che non si fosse consentito ai cittadini che lo desideravano di assistervi. Ma i cittadini erano troppi e non a tutti si sarebbe potuto concedere di farlo. Per questo, dato che allora mancavano gli strumenti per consentire l'accesso al pubblico - perché mancavano - oggi possiamo solo intuire dai verbali quale fu l'*iter* logico che consentì ai Costituenti di prendere alcune decisioni che oggi influenzano la nostra vita. Noi però abbiamo la fortuna di poter contare su mezzi e tecnologie che consentirebbero, senza provocare alcuna difficoltà, a tutti coloro che lo desiderano di assistere ai lavori comodamente da casa. Immaginate quanto ciò possa essere importante, inoltre, per uno studente universitario, delle scuole superiori oppure delle scuole medie. Immaginate Immaginate anche quale esempio si possa fornire ai cittadini e alle istituzioni di altri Paesi, mostrando la capacità delle nostre istituzioni di essere trasparenti ed efficienti. Per queste ragioni, invito sia il relatore che il Governo a modificare in senso favorevole

l'emendamento 4.107, se accolto, consentirebbe un passaggio ulteriore nella valutazione del provvedimento. Si tratterebbe di un passaggio che non allungherebbe i tempi - più di tanto - e che consentirebbe di ottenere una maggiore condivisione e diffusione nell'*iter* di approvazione. La mancata condivisione, quanto meno a livello di presidenza di Gruppi parlamentari, non escluderebbe un passaggio successivo, ma soltanto eventuale, nella parlamentari. Tuttavia, riteniamo che l'accoglimento dell'emendamento possa in definitiva rafforzare il procedimento. Nulla vieterebbe poi ai Gruppi di informare capillarmente i cittadini e l'elettorato circa quanto avviene in corso d'opera. Questo, alla luce anche dell'emendamento 4.101, illustrato precedentemente.

colleghi, l'emendamento 5.2 intende sottoporre in ogni caso al *referendum* popolare il disegno di legge o i disegni di legge costituzionale, elaborati prima dal Comitato e poi dalle Assemblee, in deroga all'articolo 138 L'emendamento proposto dal Movimento 5 stelle, in linea con i principi della Costituzione e con le richieste dei cittadini, visto che avete già bocciato fin troppe cose che tutelavano la cittadinanza, vuole maggior rispetto e intende recuperare l'elemento partecipativo che deve caratterizzare qualsiasi democrazia che voglia effettivamente definirsi tale. tale. L'approvazione di questo emendamento permetterebbe di supportare la deroga all'articolo 138 attraverso il fondamentale intervento dei cittadini elettori, accelerando peraltro, come voi volete, ulteriormente i tempi con il risparmio dei tre mesi, ovvero il tempo intercorrente tra la definitiva approvazione del presente disegno di legge e la possibile richiesta referendaria successiva. Noi chiediamo che sia a vantaggio di un vero rispetto degli elettori che ci hanno incaricato di stare qui a lavorare per loro.

a prescindere dall'utilizzo o meno di un'eventuale richiesta di un quinto dei membri della Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali prevista dalla vigente Costituzione. Colleghi, vi invito a riflettere come questo emendamento raccolga una disposizione contenuta nel disegno di legge «*quorum* zero», presentato dal Movimento 5 Stelle e a mia prima firma, che alcuni di voi sono stati propensi a sottoscrivere, estrapolando la parte di modifica del vincolo di mandato. Si tratta di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura con 50.000 firme raccolte tra i cittadini, ingiustamente ignorata da quest'Aula e mai portata in discussione: un disegno di legge che chiede con chiarezza l'incentivazione degli strumenti democratici e intende riconoscere ai cittadini anche il diritto di revisione della Costituzione. Quindi, quei cittadini si sono espressi, mediante l'*iter* previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare, di un abbassamento dei limiti del *quorum*. L'approvazione di questo emendamento, colleghi, sarebbe il primo passo verso un riconoscimento vero della sovranità popolare, segno chiaro di un processo innovatore che noi rappresentiamo e che voi spesso promettete nei salotti televisivi e nelle numerose conferenze stampa,

facendo una premessa in merito alle dichiarazioni di ieri del ministro Quagliariello, in replica ai nostri interventi e in particolare al mio intervento.

prende spunto da una mozione che è stata originata dal Parlamento. In sostanza quindi il Governo non ha fatto altro che agire a seguito di un impulso del Parlamento. Questa cosa non ce la raccontiamo! Possiamo difendere le nostre posizioni, ma sappiamo bene che quella mozione (lo abbiamo denunciato nel momento stesso in cui è stata presentata) non era altro che scritta da un Governo che aveva già un testo di legge pronto: era redatta punto per punto. Possiamo difendere le nostre posizioni in Aula, ma non ci caschiamo, signor è stato detto anche che si è passati da una Convenzione, che prevedeva esterni al Parlamento, ad un Comitato, prettamente parlamentare.

in sede di presentazione della mozione, sia dal presidente Letta in più di un'occasione, che questa riforma sarà oggetto di *referendum*. Ci è stato garantito che al popolo sarà data l'ultima parola. Eppure, nel testo del disegno di legge, malgrado abbiamo insistito in più di una occasione, in più di una occasione, è prevista ancora una volta la raccolta di 500.000 firme o di un quinto dei parlamentari di una delle due Camere: in sostanza è prevista ancora una condizione tale per cui questo *referendum*, se le maggioranze non vogliono farlo, non viene fatto.

Volevo intanto interloquire con la collega Blundo che ha illustrato l'emendamento per dire che l'opinione, che il*referendum* debba essere obbligatorio è assolutamente rispettabile:

la posizione sua e del Gruppo che rappresenta, richiama l'articolo 138 della Costituzione. Su questo punto non ci siamo. Nell'articolo 138 della Costituzione non c'è nessun *referendum* obbligatorio; anzi,

qui stiamo respingendo soprattutto gli emendamenti che non sono stati raccolti e trasformati in emendamenti della relatrice, ma questo è frutto di un lavoro che è stato fatto in Commissione, un lavoro certosino, in cui si sono raccolti molti spunti, ed è frutto anche di un lavoro che, se mi permettete, è stato fatto anche insieme ai Gruppi, tutti,

un'impostazione diversa? Delle due l'una: non si può invocare la centralità del Parlamento quando conviene e richiamare poi il Governo alle sue responsabilità quando non ci conviene più! Il testo che uscirà da questa Aula sarà quello che vorrà questo ramo del Parlamento.

il senso dell'emendamento 5.3 è molto chiaro e mi permette di motivare il voto contrario all'emendamento precedente. Noi riteniamo assolutamente opportuno che, anche con l'approvazione con una maggioranza dei due terzi delle modifiche costituzionali,

e su questo abbiamo insistito molto, anche con altri emendamenti - che le leggi costituzionali che possono essere sottoposte a *referendum*, una o più, debbano essere omogenee ed autonome dal punto di vista del contenuto e coerenti dal punto di vista sistematico. Questo perché ovviamente i quesiti devono essere molto chiari;

ne snaturerebbe assolutamente la natura. Da questo deriva anche la contrarietà alle forme obbligatorie. Ricordo sempre che

Colleghi, vi invito a riflettere. L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce che, se i progetti di legge sono approvati dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si procede comunque a *referendum*. Tuttavia questo *referendum* non sarebbe automatico, come abbiamo già visto: si può procedere alla consultazione referendaria solo se c'è la richiesta di un quinto dei membri di una Camera. L'emendamento 5.5, che abbiamo appena bocciato, intendeva garantire la nostra

nonostante l'approvazione delle leggi costituzionali avvenuta con maggioranza dei due terzi da parte di entrambe le Camere. Questo, per tutelare e rispettare le opposizioni parlamentari.

concediamoglielo: portiamole da 500.000 a 50.000, così come viene fatto per le proposte di legge popolare. Si vuole in questo caso semplificare e velocizzare la procedura - lo ripeto - e permettere ai cittadini di approvare o meno,

2», introdotto dalla Commissione, ha una finalità ben precisa. Anche in un emendamento precedente avremmo voluto eliminare la parola «elaborati», in quanto il Comitato dovrebbe, alla stregua di una qualunque Commissione (bicamerale, in questo caso), limitarsi ad esaminare i progetti di legge che gli vengono sottoposti e non elaborarne di propri.

ammetto che potrei sbagliarmi. Se mi correggerete, farò ammenda.

(forse il senatori Crimi non era presente in quella seduta). Abbiamo scritto che il Comitato «elabora» innanzi tutto in piena aderenza e coerenza con il Regolamento del Senato, che prevede che le Commissioni possano «elaborare»,

assolutamente coerente ed equilibrato, ne deriverebbe sicuramente l'esigenza, di toccare altre norme non previste nei disegni di legge originari, per mantenere l'equilibrio Questa è l'unica ragione per la quale il Comitato ha anche la possibilità di elaborare autonomamente rispetto a previsioni non contenute nei disegni di legge. Quindi non c'è alcun travolgimento dei principi che riguardano l'iniziativa legislativa: siamo in un ambito già regolato dal Regolamento del Senato, e la soluzione prevista risponde ad un'esigenza di coerenza sistematica dei testi che poi approveremo, sia in seno al Comitato che in Aula.

con l'emendamento 8.2 si intende precisare che il Comitato, fruendo di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, non abbia costi autonomi ed ulteriori, essendo composto da deputati e senatori.

dei lavori, per un richiamo al Regolamento con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 9.100. La Presidenza lo ha dichiarato inammissibile in quanto introduce una disciplina non suscettibile di applicazione per il provvedimento al nostro esame.

L'incontro ha lo scopo di chiedere al Ministro il blocco del finanziamento proveniente dai cosiddetti incentivi CIP 6, che dovrebbe ammontare a non meno di 400 milioni di euro, di soldi dei cittadini. Innanzitutto, riteniamo che oggi sia immorale privare i cittadini di tale cifra per riversarla nelle tasche del monopolista dei rifiuti Manlio Cerroni e per bruciare - con enormi danni per la salute, per l'ambiente e anche per l'economia - i rifiuti che oggi vanno considerati come una risorsa e non come un combustibile. Oltre al problema etico, esiste però un problema di legittimità: infatti i presupposti per l'accaparramento di questa cifra sono inesistenti. Sembra anche che questo magnate dell'immondizia, Manlio Cerroni, ben noto qui nel Lazio, stia facendo pressioni per una decisione *ad personam*

In tutta la questione abbiamo assistito a un *iter* fatto di scorrettezze politiche, di autorizzazioni cambiate in corsa per adattarle al ricatto, per dare alla luce un impianto firmato Termoselect,

Ancora oggi ci troviamo quindi di fronte all'urgenza di stigmatizzare un ecomostro: sarà il più grande inceneritore d'Europa e si troverà a pochi chilometri da qui, tanto per

che ha fatto andare i soldi dei cosiddetti incentivi CIP6 nelle tasche dei soliti noti: dai Moratti, responsabili del disastro Saras, a coloro che vogliono costruire gli inceneritori di Parma, di Brescia e di Malagrotta, fino allo stesso Cerroni, al quale, grazie

mi riferisco al genocidio di Srebrenica, consumatosi l'11 luglio 1995, giorno in cui oltre 8.500 uomini e ragazzi trovarono la morte nella città della Bosnia Erzegovina da cui furono deportati oltre 25.000 tra donne, bambini e anziani, il tutto di fronte all'impotenza e all'inerzia dei caschi blu dell'ONU. La memoria condivisa su una delle pagine più oscure della storia recente d'Europa rappresenta senza dubbio lo strumento attraverso cui l'Europa stessa può fare i conti con la sua storia recente, creando le basi storiche, culturali e politiche per rinnovare l'impulso dell'integrazione, in una stagione in cui le sfide e le prospettive cambiano e possono rappresentare una possibilità di rinascita per la regione. Abbiamo dunque il dovere di raccogliere l'invito dell'Europa, dando attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 2009, in cui si chiede ai Governi europei il riconoscimento ufficiale dell'11 luglio come giornata della memoria della strage di Srebrenica. Questo è un appello che rivolgo a lei, Presidente. Srebrenica è un monito per le generazioni presenti e future. Infatti le vittime di Srebrenica, e di tutte le stragi che si consumano ancora oggi in tanti Paesi del mondo, invitano a riflettere, a mettersi in discussione, a valutare in maniera opportuna il peso delle scelte che gli uomini di potere operano e che i popoli pagano. Non può esservi pace senza giustizia. E l'istituzionalizzazione di un giorno che ricorda quei momenti costituisce il modo migliore per pagare un tributo alle vittime degli orrori della storia e delineare le scelte di buonsenso del futuro.

Il motivo di questa mia accorata richiesta è dovuto ad una duplice ragione. In primo luogo, ci troviamo alla vigilia del rinnovo delle nomine dell'ente e, senza voler minimamente influenzare le prerogative dell'unico azionista di detta società, rappresentato dal Ministero dell'economia (che, peraltro, pare abbia disposto imminente convocazione dell'assemblea), sarebbe a dir poco gradita una preliminare valutazione dell'operato di detta società alla luce delle considerazioni esposte nell'atto citato. Il secondo motivo, che esula dalla specifica contingenza temporale richiamata, ma è a mio avviso perfino di maggiore urgenza, è costituito dall'insistenza con cui detta società intende riproporre l'ipotesi di istituire il pedaggio per tratte autostradali, attualmente non a pedaggio a pedaggio (come il Grande raccordo anulare, la Roma-Fiumicino, la Palermo-Catania ed altre tratte già individuate), tutte strade realizzate con risorse pubbliche. Mi permetto di insistere su questo aspetto perché, se questa ipotesi più volte reiterata dovesse prendere sostanza, come è intuitivo, essa si configurerebbe come una ulteriore tassa che graverebbe in questa particolare situazione sulla capacità di consumo e di trasferimento delle famiglie. Peraltro, l'insistenza con cui la società ne sollecita l'applicazione sarebbe finalizzata, probabilmente, a coprire i futuri disavanzi finanziari derivanti, da un lato, dall'esplosione incontrollata del contenzioso sui lavori sui lavori che si sono registrati in questi anni, pari a circa 1,3 miliardi di euro per il solo periodo 2010-2012, come si può facilmente evincere dal bilancio di esercizio della società; dall'altro lato, dal fabbisogno derivante dalle numerose perizie di variante, approvate per lo più per correggere errori progettuali commessi in passato, che hanno contribuito ad incrementare ulteriormente costi di costruzione. Basti pensare che, a fronte di 20 miliardi circa di lavori, già avviati e da avviare, l'ANAS ha a disposizione soltanto 10 milioni di euro, per compensare i futuri contenziosi e le future perizie di variante su tali lavori, con evidenti ripercussioni sulla continuità aziendale della società. La questione riveste particolare delicatezza anche in ragione di supposte ipotesi da parte della stessa società - mi sia passato il termine un po' grossolano - di fuoriuscita dal perimetro della pubblica amministrazione, proprio in ragione della natura di tali cespiti, che non sono più inquadrabili come trasferimento di risorse pubbliche. Presidente, io sono certo di confidare, oltre che nella vostra sensibilità e attenzione per la problematica che ho posto, anche nella consapevolezza da parte del Governo della delicatezza delle questioni e voglio pertanto supporre che questa mia richiesta e l'auspicato vostro interessamento possano consentire di ottenere le risposte richieste con l'atto ispettivo in questione. Lo dico

Nello stabilimento chimico dell'ICMESA una valvola di sicurezza del reattore A-101 esplode, provocando la fuoriuscita di alcuni chili di diossina nebulizzata (TCDD), la più pericolosa delle diossine ed oggi volgarmente conosciuta proprio con il nome di «diossina Seveso». Per cinque lunghi giorni i tecnici dell'ICMESA e le autorità rassicurarono e minimizzarono. Solo dopo una moria diffusa di animali e piante ed altri casi di intossicazione, viene emanata un'ordinanza: divieto di toccare la terra, gli ortaggi, l'erba, di consumare frutta, verdura, animali da cortile e di esporsi all'aria aperta; si consiglia un'accurata igiene della persona e dell'abbigliamento. La nube tossica interessa il territorio di sette comuni (Meda, Barlassina, Seveso, Seregno, Cesano Maderno, Bovisio, Desio) e una popolazione di circa 100.000 persone. I casi di intossicazione aumentano e i più colpiti sono i bambini. Si dà il nome ad una malattia finora quasi sconosciuta: la cloracne. Un numero imprecisato di bambini rimane sfigurato dalla cloracne e porterà per sempre sulla propria pelle gli effetti di questa micidiale sostanza. I danni sanitari, materiali e morali di questo disastro ecologico provocato dall'uomo restano incalcolabili. anni di distanza da questo disastro, il terreno è ancora intriso di diossina. Nonostante lo stabilimento chimico sia stato interrato e al suo posto ci sia ora il Bosco delle querce, impiantato nella zona a segnare, con un itinerario nella memoria, un evento da non dimenticare, lo Stato sembra invece aver dimenticato e oggi progetta un'autostrada, la Pedemontana, che violerà proprio il Bosco delle querce e interverrà con cantieri e movimento terra proprio nelle aree contaminate. Il Movimento 5 Stelle non dimentica. E non dimentica che oggi il territorio italiano conta circa mille aziende a rischio di incidente rilevante, molte delle quali insistono in aree fortemente antropizzate, mettendo a rischio la vita di centinaia di migliaia di persone ipotecando negativamente lo sviluppo sostenibile di città e territori dall'inestimabile valore ambientale, storico e culturale.

Questa notte c'è stato un ennesimo attacco militare (non c'è bisogno che lo illustri, perché i giornali ne stanno parlando in modo molto approfondito) da parte di una cinquantina di incappucciati, che hanno attaccato le forze dell'ordine a Chiomonte e gli operai che lavoravano per il terzo turno con bombe carta e un mortaio che sparava bengala ad altezza uomo. Ci sono le foto che illustrano perfettamente tutto l'attacco e credo che tra qualche ora la stessa questura di Torino metterà a disposizione i filmati. disposizione i filmati. Il collega Scibona leggeva la lettera di una cittadina in cui si parlava di «strani incidenti, mezzi che si incendiano, operai che vanno al pronto soccorso. Tante storie da verificare, ma regolarmente assegnate alla violenza scatenata dai "no Non so dove viva la cittadina che ha scritto la lettera al collega Scibona, ma so come vivono ormai da due anni gli operai, i tecnici, i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri in quel cantiere. Ho sostenuto in questi anni una battaglia politica a difesa della Torino-Lione, però, se devo devo mettere in conto che lo Stato non è in grado di fermare cinquanta delinquenti che hanno l'unico scopo di far male e di uccidere, credo che a questo punto si possa tristemente prendere prendere atto che la legalità e la democrazia sono sconfitte. Ritengo che mettere a rischio la vita di persone che lavorano, sperando che la fortuna ci aiuti sempre, non sia degno di uno Stato democratico.